non sono puniti in maniera fine a se stessa ma quando dall'incitamento, istigazione o propaganda derivi un concreto pericolo di diffusione - e quindi il rischio concreto che si possa determinare la commissione di un delitto

peraltro in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ma anche con la giurisprudenza della Corte costituzionale, e non soltanto in materia di reati di pericolo e di reati di opinione. Ci troviamo, infatti, nel tema caldo

tale. L'espressione pertanto trova anche conforto nella giurisprudenza di legittimità e nella giurisprudenza costituzionale che riconoscono il delitto di opinione compatibile con il nostro assetto costituzionale se effettivamente determina un concreto pericolo che qualcosa ne possa derivare.

però di un termine che, in un certo senso, non rende l'idea completa della garanzia che si deve soddisfare sul punto. Analogamente, si tratta di un termine anacronistico. Quindi non è vero che tra pubblico e privato non ci siano situazioni in fatto, soprattutto determinate dalla modernità, che non meritino di essere prese in considerazione. Cosa intendo dire? Perché questa espressione è più garantista del termine «pubblicamente»? La circostanza che un fatto venga commesso in pubblico determina soltanto una presunzione di diffusione dell'incitazione, dell'istigazione o della propaganda perché taluno in una piazza, a ora notturna, può compiere operazioni di incitamento o istigazione senza che nessuno lo ascolti e, quindi, senza che vi sia il rischio di un propagarsi e di una diffusione dell'incitamento. Quando si utilizza il termine «pubblicamente» si evoca una categoria importante - lo riconosco in maniera assolutamente chiara - che però non risolve integralmente il problema per come, al contrario, lo risolve meglio un'espressione che fotografa ciò che dal «pubblicamente» dovrebbe derivare, ossia un pericolo concreto di diffusione dell'istigazione, dell'incitamento o della propaganda. che l'espressione «pubblicamente» è anacronistica perché rappresenta, in un certo senso, il conflitto tra il pubblico e il privato, tipico di una società che non conosceva il mondo dei *social network* e del *web*. infatti contesti della modernità che, pur sfuggendo alla definizione e all'etichetta pubblico o privato, possono determinare la diffusione incontrollata e quantitativamente drammatica di fatti che costituiscono incitamento all'odio, alla violenza e quant'altro. L'espressione «pubblicamente» non copre quest'area

telematici, si concretizzerebbe in fatti che - ripeto - non sono pubblici (chi scrive all'interno della propria stanza su un sito diffondendo proclami terroristici non lo fa certamente in pubblico),

che non si punisce il negazionismo della Shoah, dei crimini di guerra, di genocidio e contro l'umanità fine a se stesso, così determinando il rischio di impedire il dibattito culturale. Ciò

la Shoah e i crimini di guerra, di genocidio e contro l'umanità per incitare alla violenza. Questo è l'assetto della norma. Quindi, se taluno si limita a negare, ma non funzionalmente, cioè strumentalizzando la negazione per incitare alla violenza, il fatto non è di rilevanza penale. Per tali motivi, ritengo che l'emendamento 1.401 risolva il problema di una punibilità estesa a fatti che non possono definirsi pubblici

e la pubblicizzazione, come sapete, è collegata alla "legge Mancino" e a un'aggravante che scatta quando ci sono motivi etnici o razziali. È una bestialità: diamo l'aggravante a chi nega alcuni avvenimenti. In realtà, sono centinaia di avvenimenti. Ho scritto ieri un articolo: si va dalla vicenda degli indiani d'America, alle attuali vicende di Israele, alle guerre in Bosnia, alla vicenda coloniale italiana. Infatti, secondo questo disegno di legge, tutto il dibattito fra Indro Montanelli e Del Boca sulla nostra vicenda coloniale - in cui Del Boca sosteneva che l'Italia avesse compiuto atti di genocidio e crimini di guerra e Montanelli lo negava,

chi pubblica un libro in cui esprime una visione di un certo tipo della nostra vicenda coloniale. Ma la bestialità è che noi colpiamo con un'aggravante chi nega il genocidio, la Shoah, i crimini di guerra, ma non chi li esalta. Infatti, se io nego il genocidio armeno ho l'aggravante; se lo esalto, dicendo che hanno fatto benissimo, non ho l'aggravante.

poi, che questo testo riguarda migliaia e migliaia di casi. Amici di Israele - e ce ne sono - vi prego di andare a leggere sui siti le dichiarazioni del Governo iraniano,

sulla razza e sull'etnia. Si dice che a Gaza, nel momento in cui Israele si è difeso, per ragioni razziali ed etniche (esattamente quelle che noi abbiamo previsto nel nostro disegno di legge), ha compiuto crimini di guerra.

io scriva un libro negando che Israele sia un Paese razzista o che agisca per ragioni di pulizia etnica, come i suoi avversari e come i Governi ammettiamo che io neghi l'esistenza di questi crimini di guerra; che cosa succede? Che ho l'aggravante punibile con la reclusione da due a sei anni? Certo, l'obiezione in Commissione è stata: ma poi al processo te la cavi. Arriverà la denuncia, ma poi si andrà vedere il limite e la propaganda che è stata fatta di determinati avvenimenti, che riguardano Israele. Io l'ho detto che la vera vittima di questa legge si chiama Stato di Israele.

Andate a vedere i crimini di guerra: 170 criminali di guerra bosniaci, croati, serbi, già condannati da un tribunale internazionale in una guerra che è stata di pulizia etnica di serbi contro croati, croati contro serbi, musulmani contro cattolici croati. In tutti i singoli e terribili episodi di quella guerra,

stabilire che un determinato episodio lo nego perché lo attribuisco non ai croati ma ai bosniaci, oppure non ai bosniaci ma ai serbi? Oppure la mia è una propaganda a favore della pulizia etnica, nel momento in cui non corrispondo a una visione di parte? Parliamo dello sterminio degli indiani d'America. C'è un termine tecnico che lo indica, ma posso sostenere che era inevitabile e non che fosse un genocidio, come viene chiamato, perché sono arrivate dall'Europa persone che avevano una cultura un modo di operare tecnico molto superiore a persone che erano rimaste sostanzialmente al neolitico. Oggi ci sono 300 milioni di persone negli Stati Uniti e c'era un milione di nativi. Posso dire che c'era una superiorità etnica dei bianchi quando sono andati in America rispetto ai nativi e che tutto ciò ha determinato una situazione che contesto essere stata un genocidio? No, perché mi si applica l'aggravante. Io per questa affermazione posso essere denunciato, per il combinato disposto della legge Mancino e di quello che abbiamo scritto. Se quest'Aula, come al solito, vuole fare finta di niente, quando il prodotto legislativo uscirà riceverà fischi, lazzi e pernacchie da tutto il mondo del diritto e degli storici, e verrà preso come una stravaganza.

vostra moglie o un parente avvocato vi domanderanno «scusate, ma voi oggi che reato o che aggravante avete applicato?» provate a spiegare loro che il Parlamento ha approvato un'aggravante e provate a spiegare il combinato disposto dell'articolo 3 della legge Mancino

crimini di guerra: la «distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari»; la «deportazione, trasferimento o detenzione illegale»;

Questi sono crimini di guerra. Come si fa in operazioni militari, ad esempio di autodifesa, come quelle di Israele, a stabilire che queste fattispecie, che sono fisiologiche quando c'è un conflitto, sono crimini di guerra

quando si nega una certa circostanza delle migliaia che ho citato o una storia come quella coloniale italiana, o la storia degli Stati Uniti o quella di Israele o quella della guerra dei Balcani e contemporaneamente invece non condanniamo chi esalta

non si sapeva a quale scopo recondito mirassi. Invece, affinché tutti lo sappiano, tale emendamento era stato presentato dalla relatrice, a cui do atto

perché lei mi insegna che la legge n. 654 del 1975 fu modificata dall'onorevole Mancino nel 1993

il presidente Zanda, con il quale ci conosciamo da anni, mi invitasse a casa sua e io lì parlassi

Avevamo introdotto un equilibrio, che il codice penale pretende, in ragione dell'istigazione: un equilibrio tra la libertà di espressione di qualsiasi idea e l'ipotesi del reato che deve essere tale da incidere e, quindi, ecco le ragioni del «pubblicamente». Allo stesso tempo ci avevano detto, in particolare il Governo, il testo era stato modificato in Assemblea perché si erano preoccupati dell'ipotesi del terrorismo. Allora, rispetto al testo votato dal Senato, il mio emendamento prevedeva un aggravante specifica per l'ipotesi del terrorismo, tenendo conto proprio delle indicazioni venute dal Governo e dalla maggioranza. Improvvisamente siamo usciti dalla Commissione che sul punto del «pubblicamente», afferente alla prima parte

il Governo chiedeva di trovare una soluzione che potesse tener conto del mio emendamento. Ma sulla prima parte, che avevamo già votato tutti all'unanimità, non c'era stata discussione. E allora che è successo?

perché condannava certe espressioni che politicamente sono ancora presenti nel nostro Paese. Credo che avrebbe avuto una diversa forza.

Non ho alcuna intenzione di dilazionare i tempi di approvazione di questo disegno di legge, però registro, sia pur in piccolo, il persistere di una prassi che da ultimo la Presidenza del Senato ha stigmatizzato

di attenzione. È chiaro che con questo emendamento è preclusa ogni forma di discussione su tutti gli altri emendamenti. Sostanzialmente non sarà possibile trattare i singoli temi

rispetto a un emendamento che singolarmente viene presentato dal Presidente e non dal relatore del provvedimento stesso. Però, ormai le cose sono fatte e gli accordi sono raggiunti, per cui comprendiamo perfettamente quale sarà l'esito del percorso successivo. poiché vorremmo intervenire prima che si metta in votazione l'emendamento 1.401, vorremmo avere la certezza che ciò ci sarà consentito. Senatore Palma, la Presidenza è consapevole di quello che lei ha detto, tant'è che

ancora espressi - alle dichiarazioni di voto finali, che quindi consentirebbero all'Assemblea di pronunciarsi anche sulla proposta innovativa, che diventa di per sé il disegno di legge. Però noi avremo anche la possibilità di intervenire nella discussione sull'articolo 1. Quindi, è possibile intervenire prima ancora di questa fase delle dichiarazioni di voto finali. L'eventuale approvazione dell'emendamento 1.401 porterebbe all'approvazione del disegno di legge nel suo complesso. Quindi, è ovvio che la sua domanda sulla preclusione

Quindi, per essere chiari, signor Presidente, avendo io non piccole perplessità in ordine all'emendamento 1.401 e avendo intenzione di intervenire su questo in termini critici e più specifici rispetto all'intervento del senatore Caliendo, quand'è che mi sarà consentito intervenire? Prima della votazione o no? Se non è prima della votazione, chiedo di intervenire nella fase dell'illustrazione degli emendamenti avendo io presentato un altro emendamento.

Adesso possiamo fare la discussione sull'articolo 1 e, quindi, i colleghi possono intervenire. Il senatore Quagliariello si sta iscrivendo a parlare. Abbiamo la richiesta sua e dei senatori Malan,

in questo caso la questione sia ancora più grave, perché il firmatario dell'emendamento è il Presidente della Commissione giustizia e, quindi, ci sarebbero stati tutto il tempo e la possibilità per poterne discutere in Commissione.

approvati dall'Assemblea. In particolare, l'ultimo periodo di tale comma dice che «il Presidente può tuttavia consentire, quando se ne manifesti l'opportunità, la presentazione di emendamenti al di fuori dei casi anzidetti». momento che credo si tratti di una situazione di assoluta eccezionalità, che rischia di creare una prassi che impedisce al Parlamento di votare tutti gli altri emendamenti, le chiedo di disporre di un'ora di tempo per poter presentare i subemendamenti all'emendamento D'Ascola

finestra"). Comunico che i fogli recanti le firme per la richiesta di *referendum* popolare, promossa da un quinto dei componenti del Senato, sul testo di legge costituzionale recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione», sono stati consegnati, su richiesta dello stesso, al senatore Luigi Zanda, delegato, con i senatori Renato Schifani e Karl Zeller, a depositare la richiesta presso la cancelleria della Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

servite le dichiarazioni avventate di qualche parlamentare dell'altro ramo del Parlamento. Il problema che si pone Il problema che si pone riguarda principi importanti quali la libertà di opinione e di manifestazione del pensiero. Come sempre accade, il tutto viene buttato in confusione. Il termine «pubblicamente» avrebbe l'effetto di far venire meno tutta una serie di processi penali pendenti per i reati di cui all'articolo 3 della legge n. 654 del Quanti e quali sono questi processi? Ahimè, dispiace dover dire che non vi è traccia di questi processi pendenti. Quindi, sostanzialmente, siamo in presenza di una suggestione che si ancora al nulla. Ho letto con attenzione l'emendamento presentato non dalla relatrice, ma dal presidente D'Ascola, così come con attenzione ho ascoltato il suo intervento. Devo dire la verità: non mi sembra che il presidente D'Ascola abbia fatto un grande sforzo di carattere teorico o dottrinario. Nel momento in cui propone di sostituire la parola «pubblicamente»

del 1975, in virtù della quale si afferma che non ogni istigazione pubblica viene punita, ma deve essere punita quella istigazione pubblica che, per le sue modalità, sia in grado di cagionare un concreto pericolo di diffusione. Quindi - mi scuserà il presidente D'Ascola - vi è una corretta opera compilativa e non vi è alcuna opera di carattere creativo. Ho altresì ascoltato, nell'intervento del presidente D'Ascola, che vi sono altre modalità di istigazione o di incitamento, faceva riferimento - ad esempio - a Facebook e sostanzialmente ai mezzi informatici. Ma ricordo al presidente D'Ascola che l'articolo 414, quarto comma, prevede, per l'appunto, un ulteriore aggravamento di pena proprio quando l'istigazione (in quel caso) viene commessa attraverso i mezzi informatici. Quindi, le modalità del mezzo possono costituire un'aggravante, ma non portano acqua al mulino dell'obiettivo percorso. La verità di fondo, signori senatori, è che in Commissione giustizia si era raggiunto un accordo pieno sul testo del provvedimento. Ma poi - chissà perché - il convitato di pietra presente in quest'Aula (anche se non si vede) ha dato un *input* diverso e, attaccando il senatore Caliendo, ha richiamato all'ordine i componenti del suo partito facenti parte della Commissione: non vi può più essere il termine «pubblicamente». Ma se non vi può più essere il termine «pubblicamente», signori senatori, che senso ha scrivere «cagioni il concreto pericolo di» se questa è la formula che la Corte costituzionale indica per concretizzare l'istigazione pubblica? Si tratta di un emendamento ipocrita, che cerca sostanzialmente di salvare capra e cavoli, di lasciare intatto il concetto del «pubblicamente», evidentemente sostituendolo con le parole della Corte costituzionale.

alla lettera *a)* si prevede una pena fino a un anno e sei mesi per determinati comportamenti e alla lettera *b)* si prevede una pena fino a quattro anni per altri comportamenti. In entrambi i casi vi è il termine «istiga». Vi rendete conto che, nel momento in cui, seguendo l'emendamento del senatore D'Ascola, inseriamo un nuovo comma e diciamo che, se i comportamenti di cui alle lettere *a)* e vengono posti in essere in modo tale da cagionare un concreto pericolo, fondandosi sulla Shoah o sulla negazione di altri crimini di guerra, automaticamente si afferma la punibilità delle lettere *a)* e *b)* normale, cioè dell'ipotesi base, anche quando l'istigazione non è tale da cagionare un concreto pericolo? Il che equivale a dire - per quanto possa essere spiacevole e assolutamente intollerabile la frase - che se nella vostra vita privata (ad esempio

in totale eccezione rispetto al sistema, che prevede la punibilità dell'istigazione solo se accolta - e in quel caso vi è un concorso nel reato commesso - o la possibilità per il giudice di irrogare una misura di sicurezza ove non accolta.

sostanzialmente il legislatore correttamente punisce non l'istigazione di per sé, ma il pericolo che può derivare da un'istigazione pubblica e, quindi, lesiva del cosiddetto ordine pubblico. Ma sotto questo profilo affronteremo, poi, con riferimento ai singoli punti le perplessità che io ho avuto. Mi permetto di dire una cosa. La lettera *a)* dell'articolo 3 della legge Reale punisce un determinato comportamento (propagandare la superiorità, l'odio razziale e via dicendo) con una pena fino a un anno e sei mesi punisce con una pena fino a quattro mesi chi invece istiga o commette atti di violenza. Mi spiegate la ragione per la quale due comportamenti puniti dal legislatore in termini diversi, perché diversa è la loro gravità, devono avere una punizione identica in ragione dell'emendamento D'Ascola? E per quale ragione - ad esempio - il comportamento previsto dalla lettera che è punito fino a un anno e sei mesi di massima, dovrebbe essere punito fino a sei anni, cioè con una pena tre volte superiore il suo massimo? E come non potete non vedere che la pena fino a sei anni per chi propaganda l'odio razziale fondandosi sulla negazione della Shoah Shoah è nel minimo superiore e nel massimo di poco inferiore a chi istiga pubblicamente la commissione di delitti di terrorismo?

che il sistema penale non consente distonie irragionevoli, salvo l'intervento della Corte costituzionale. Ed è per questo che noi avevamo inserito il termine «pubblicamente» prima e avevamo di poco abbassato, nel totale accordo di tutti, i massimi di pena previsti per il reato di istigazione a commettere delitti. Come ultimo punto,

se la propaganda si fonda sulla negazione della Shoah. Mi spiegate voi la ragione per la quale,

per gli storici, per qualche pazzo di passaggio negare la Shoah. Ma mi spiegate la ragione per la quale, se io commetto tutta una serie di comportamenti senza negare la Shoah,

effetti, mentre non può essere punito nello stesso identico caso, cioè un'istigazione non produttiva di effetti, se dice la stessa identifica cosa fondando, però, il suo dire sulla negazione della Shoah. È materia semplice, è materia di buon senso. Come non vi rendete conto che questa legge, che accontenterà il convitato di pietra, sostanzialmente presta il fianco

perché parliamo di un provvedimento importante al quale diamo molto rilievo e che ha come oggetto la speciale punibilità per comportamenti di negazione di un

tempo per subemendare un testo di origine parlamentare, dico che non ricordo grandi precedenti in cui questo tempo sia stato concesso e abbia prodotto 17 subemendamenti.

e personalmente a ciascun senatore. Teniamo conto di cosa stiamo discutendo. Stiamo discutendo di una cosa molto seria e delicata. Io personalmente sento un dovere.

riprendo logicamente quello che ci ha comunicato il presidente Zanda. Egli ci ha detto che in Commissione è stato svolto eccellente e approfondito; ne ha dato atto al senatore Caliendo. A questo lavoro ovviamente hanno partecipato i membri della Commissione, Commissione, tuttavia esso è stato fondamentalmente smentito da un emendamento presentato direttamente in Aula. Io ho ascoltato il dibattito che ha introdotto la giornata di oggi; se non ho compreso male le parole del collega Caliendo, lui ritiene che quel lavoro sia stato oggettivamente smentito. Questa dinamica si innesta su una situazione di fatto, senatore Zanda, sulla quale vorrei poi tornare nel corso del dibattito, ma che vorrei fosse chiara già in partenza: qui non è un dibattito tra chi ritenga che la Shoah non sia stata un crimine orribile e chi ritiene invece che lo sia stata.

prescinde da quanto è stato fatto in Commissione e richiede un approfondimento in quest'Aula: il problema è se su temi di questo tipo sia possibile introdurre reati di opinione, ovvero se questi appartengono, anche quando colpiscono fattispecie come quelle di cui stiamo parlando, parlando, a una cultura non liberale, di cui abbiamo una traccia profonda in un codice che risale a un altro periodo della nostra storia, e pertanto vanno trattati con moltissima attenzione.

intervenire nel merito, ritengo che non ci debba essere alcun atteggiamento ostruzionistico,

nella interazione tra Commissione e Aula, né tanto meno dalla profondità della materia, perché come intervenire su questa materia è argomento sul quale in altri periodi sono stati spesi dibattiti parlamentari che sono durati mesi e mesi. Francamente se si spende qualche momento in più per discutere qualche subemendamento che è stato prodotto in una sosta di tre quarti d'ora non credo che sia un crimine e nemmeno una lesa maestà.

aprire un minimo di discussione su questi subemendamenti a un emendamento che travolge completamente il lavoro fatto in Commissione. Credo che questo sia un appunto che non possa essere accettato o forse nemmeno tollerato. il lavoro che è stato fatto in Commissione, peraltro raggiungendo ampi margini di maggioranza se non quasi di unanimità, al fine di dare un equilibrio all'intero sistema e riconoscendo che la legge Mancino desta talune perplessità,

può ritenersi più abile o più efficiente di qualsiasi altro, si incorrerebbe in un crimine. Ritenevamo che la legge Mancino fosse di per sé mal strutturata e necessitasse di un intervento e ciò che avevamo fatto in Commissione era un lavoro giusto.

Sono perfettamente d'accordo nel colpire la negazione di un fatto storico di una gravità mai vissuta nella storia dell'umanità come l'olocausto del popolo ebraico.

persona, mi sembra incredibile. Come facciamo a mettere nello stesso testo e punire con la stessa gravità di sanzione chi nega l'olocausto e chi nega una delle 20.000 fattispecie che sono già dinanzi ai tribunali internazionali in tutto il mondo, dalle guerre balcaniche

che si applica la reclusione da due a sei anni se «la propaganda» viene commessa «in modo che derivi concreto pericolo di diffusione». Ma la propaganda, se prendete qualsiasi dizionario, significa diffondere e divulgare. Si colpisce la propaganda se c'è il pericolo concreto che la propaganda venga diffusa? Si può scrivere per legge una cosa di questo genere, quando la propaganda per definizione è diffusione di qualcosa? È come dire che è lecito scrivere un articolo o un libro in

ha stabilito per legge che quello del popolo armeno è stata un genocidio; la Turchia, per legge, manda in galera chi dice che quello del popolo armeno è stato un genocidio. È un caso concreto di genocidio su cui due Paesi si sono scontrati: è un grande problema internazionale e c'è un grande dibattito. La Turchia può entrare in Europa, se nega quello che è accaduto? Ma se queste cose fondamentali, come l'olocausto e il genocidio, le annacquiamo tra decine di migliaia di casi, ognuno dei quali diventa oggetto della legge

ieri - e lo ridico oggi - che in queste norme vedo la concreta possibilità che l'unica vittima di questa normativa siano proprio Israele e il popolo ebraico, con l'interpretazione che verrà data al testo così come l'abbiamo scritto. Il Senato aveva trovato delle formule comunque giuridicamente soddisfacenti, ora pensiamo di approvare una norma che si sottopone non alla critica, ma al ridicolo, perché questa storia della propaganda

Quali processi sono attualmente in corso per la violazione della legge Mancino? Dove sono le decine di processi e le persone che dovrebbero farla franca rispetto alla violazione della legge Mancino? Dove sono?

che si sarebbero dati da fare per togliere, all'interno dei processi, la giusta condanna a chi aveva violato la legge Mancino e stamattina qui nessuno è in grado di dire se vi sia una persona che sia oggi sotto processo. Noi, invece, se approviamo questo testo, intendiamo correre il rischio di mettere sotto processo decine di persone che esercitano semplicemente il loro diritto di propagandare delle idee.

che l'abbattimento di case durante un'operazione di guerra abbia la stessa pena, nelle fattispecie che abbiamo indicato, dell'olocausto. Come facciamo a mettere sullo stesso piano la più grande tragedia dell'umanità con altre mille fattispecie? fattispecie? Credo che tornare in Commissione, rivedere il provvedimento e riportare un testo unitario sia la cosa più saggia che possiamo fare, anche per non essere in contraddizione con noi stessi, con un Senato che qualche mese fa aveva votato all'unanimità un testo che oggi viene stravolto.

Grazie,

Presidente, mi consenta una breve replica, che mi ero riservata di svolgere dopo l'illustrazione degli emendamenti e dei subemendamenti. Si tratta di un provvedimento che giunge in Senato in terza lettura e che ha visto confrontarsi due proposte di intervento diverse, direi opposte, tra la Camera e il Senato.

ci siamo chiesti se ci fosse la possibilità di individuare un ambito di intervento che fosse un ambito ambito mediano tra quello che è stato individuato alla Camera e quello che è stato individuato al Senato. Il Governo si era rimesso alla Commissione ed aveva auspicato un'ulteriore riflessione, che giunge in quest'Aula con la proposta del senatore D'Ascola, sulla quale il Governo esprime parere favorevole. In Commissione e poi di nuovo qui in Assemblea, il senatore Caliendo in particolare ed in Aula oggi, con grande puntualità, anche il senatore Nitto Palma hanno posto un altro tema, che però esula dal contenuto contenuto stringente di questo intervento legislativo: l'armonizzazione delle pene sui reati di istigazione. Il Governo raccoglie questo invito alla riflessione e si dichiara disponibile ad approfondire questo tema.

Tuttavia dopo aver ascoltato il senatore Zanda, e soprattutto dopo avere ascoltato il compromesso sul compromesso del compromesso che ci è stato proposto dal sottosegretario

le altre cose, di produrre effetti assolutamente opposti a quelli che si prefigge: Popper le avrebbe chiamate conseguenze inintenzionali. E poiché è proprio alle più giuste delle battaglie di merito che si fa maggior torto se le si combatte con un metodo sbagliato, vorrei che ci sforzassimo di separare i piani. Per questo dico che è tanto più un dovere opporsi a questo disegno di legge, e chiedere che sia integralmente soppresso, quanto più si considerano ignobili e aberranti le teorie che si intende mettere fuori legge. Su questo la mia opinione è anche più estrema di quella del collega Giovanardi: per quanto mi riguarda non c'è nemmeno da operare una distinzione tra la Shoah e le altre fattispecie.

Shoah, abietta, ridicola e insostenibile sul terreno del confronto logico-storico. Coloro che se ne fanno portatori sono oggettivamente dalla parte del torto. mettere le opinioni fuori legge non è la strada giusta per contrastare i cattivi pensieri; anzi, è vero il contrario. Al di là delle contraddizioni e delle aporie insite nel testo in discussione, che si innesta su una legge che sarebbe essa stessa da riconsiderare, la legge Mancino; al di là del balletto su una modifica che quantomeno avrebbe attutito i rischi; al di là della vaghezza di una formulazione che, riferendosi genericamente al genocidio, ai crimini di guerra, ai crimini contro l'umanità, investirebbe non solo la storiografia ma anche il dibattito sulla geopolitica attuale,

vi sono a mio avviso, signor Presidente, ragioni di fondo per opporsi a questo disegno di legge. Innanzi tutto una contrarietà di principio al reato di opinione, anche l'opinione più aberrante, come in questo caso. L'opinione non è un reato, mai. E la storia ci insegna che contrastare i cattivi pensieri comprimendo la libertà è il modo migliore per alimentarli. Diverso è il caso della diffamazione; diverso, ovviamente, è il caso dall'incitamento a delinquere o a commettere concretamente atti di discriminazione per motivi razziali, civili, nazionali o religiosi. Ma qui ci troviamo in altri ambiti del diritto penale che sarebbe bene non confondere con la sfera delle opinioni, che al dritto penale io credo debbano rimanere totalmente estranee. Le opinioni si combattono con le altre opinioni; si combattono nelle aule delle scuole, delle università, non in quelle dei tribunali. Si combattono con le parole, con i mezzi di diffusione delle stesse; si combattono con la cultura, con l'esempio, con la memoria e con l'educazione. Non si combattono con la galera, mai. In secondo luogo, nelle maglie di norme di questo tipo, soggette ad ampia discrezionalità interpretativa, le migliori intenzioni del legislatore

vi sono opinioni che rimuovono o anche giustificano il genocidio e i crimini contro l'umanità perpetrati dal regime comunista: quelle pagine nei manuali di storia e non le condivido, ma non vorrei mai che fossero catalogate come reato. Infine - ed è un tema che come legislatori ci interpella direttamente - credo che il disegno di legge in esame si inscriva in una più generale tendenza a credere che con lo strumento penale si possano risolvere tutti i mali della società. Non è così e, così facendo, stiamo progressivamente distorcendo la natura stessa del diritto penale. Signora Presidente, colleghi, trovo molto preoccupante che il legislatore tenga sempre meno conto del principio di tassatività delle norme incriminatrici che scaturisce dal nostro ordinamento costituzionale. E sfido chiunque a dimostrare cosa ci sia di tassativo nel provvedimento in esame che a tutti gli effetti è una legge bandiera, destinata nel migliore dei casi a restare disapplicata e, nel peggiore, a produrre assurdità. Se tutto è penale, alla fine nulla sarà penale. È difficile pretendere più sentenze in tempi più rapidi e capi d'accusa

dall'autocertificazione per il canone Rai alle opinioni, per sballate che siano, sulla storia e sull'attualità. Signora Presidente, non ce la prendiamo poi con i magistrati se produciamo leggi di questo tipo. In un'Assemblea in tutti si dicono liberali è forse bene che un'opinione come questa, per quanto minoritaria e per quanto l'emendamento in esame sia destinato a essere sconfitto, entri e si faccia sentire.

però segnalare, sulla base di quello che ha detto l'esponente del Governo, una sgradevole e sguaiata mancanza di rispetto nei confronti del nostro Gruppo avvenuta nelle ultime quarantott'ore in Senato.

non solo per la serietà, collega Zanda, ma anche per l'onestà di intenti con cui si era lavorato in Commissione. Tutto era incentrato sulle benemerenze del termine «pubblicamente».

del dibattito a cui aveva partecipato in Senato, ma su un'intervista della Presidente della Commissione giustizia della Camera dei

il senatore Liuzzi, in quanto membro della Commissione 7a e non della Commissione giustizia, non sia stato minimamente avvisato. Meno ancora è stato avvisato - e non posso credere alla sua mancanza di buona fede

emendamento. Lo stesso sento che è capitato alla senatrice Stefani. Ecco, allora, quello che volevo dire prima sull'ordine dei lavori: non è la prima volta che capita. di un Gruppo, di un partito, quello di maggioranza, ma queste non cancellano, almeno sul piano dell'informazione, le prerogative dell'Assemblea.

- si riaprisse una discussione. Ma siamo seri! Alcuni colleghi hanno proposto come subemendamento, invece che «in concreto pericolo» soltanto «in pericolo». Io non metto in dubbio che il senatore D'Ascola sia un grande compilatore e non lo dico nel senso denigratorio al quale forse alludeva il collega Palma; se, però, non ci fosse mai stato il «pubblicamente» e fossimo partiti dalla formulazione «propaganda con concreto pericolo di diffusione», probabilmente un minimo di discussione parlamentare ci avrebbe fatto approdare al «pubblicamente». La verità è che in questo provvedimento ci sono molte, molte ipocrisie; non la nostra e di nessuno del nostro Gruppo e se il collega Zanda ci volesse invitare, insieme a Caliendo, a casa sua, stia tranquillo che nessuno di noi dirà bestemmie sulla non esistenza della Shoah. Ma l'utilizzazione della giurisdizione internazionale per delegittimare lo Stato di Israele è un movimento politico: si chiama BDS, opera a Ginevra e alle Nazioni Unite, forse è una vecchia idea di un vecchio segretario delle Nazioni Unite, Waldheim (il nome dovrebbe dire qualcosa). Ecco le ragioni per le quali abbiamo molte difficoltà a non votare per gli emendamenti. Sul voto del provvedimento mi pronunzierò in sede di dichiarazione di voto finale. Comunque rimpiangiamo, senatore Zanda, quel grande Paese, gli Stati Uniti d'America, dove approvare una legge contro la libertà d'opinione non solo preclude i voltairismi ben calibrati dell'amico Quagliariello, ma è una garanzia in sé di incostituzionalità. Invece qui si è sostituito il «pubblicamente» con una ginnastica lessicale - dico bene, collega Palma? - ricavata da una precedente sentenza della Corte costituzionale. Di qui il nostro voto a favore dell'emendamento. non so quale sarà l'orientamento del mio Gruppo, ma su queste tematiche che hanno un valore inestimabile e che riguardano la libertà di espressione e di opinione di una Nazione ritengo che non ci possano essere vincoli di alcun tipo. Sottoscrivo appieno quello che ha testé

noi avremmo propagandato, nel senso più nobile del termine, quelle idee e quegli avvenimenti

ha ragione, perché in uno Stato di diritto, in uno Stato libero, vale la massima di Voltaire: «Signori, non sono affatto d'accordo con quello che dite, ma darei la mia vita perché voi possiate continuare a dirlo». Questa legge non serve a niente, se non a mettere un ulteriore ulteriore grimaldello nelle mani dell'unico potere che esiste in Italia inconferente ed irresponsabile, il potere della magistratura, Grazie,

e fino a quando non vi sarà la nuova legislatura con l'Italicum, questo, sia pur in termini desueti, si chiama tuttora Parlamento e non "zittamento". Con la conseguenza, senatore Zanda, che lei e i suoi colleghi dovete usare la pazienza di ascoltarci; e il parlare non sempre si ispira a fini ostruzionistici. Senatore Zanda, prendo atto con favore che non è suo costume adeguarsi ai desideri dei convitati di pietra; non l'avevo detto, e le ricordo il detto sull'*excusatio non petita*. Sicuramente, come lei mi ha accusato, non è mio costume seguire i *Diktat* dei convitati di pietra: se ho un difetto, è quello di fare a viso aperto tutto quello che ritengo di dover fare. Signori senatori, il discorso è molto semplice e vi chiedo un attimo di attenzione. L'articolo 3

o con la multa fino a 6.000 euro chi istiga a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Il che equivale dire che se io istigassi il senatore Caliendo ad uccidere il senatore Malan non incorrerei in alcuna pena se il senatore Caliendo, evidentemente, avesse la bontà di non accogliere l'istigazione. Ciò perché il nostro codice penale, all'articolo 115, impedisce la punibilità dell'istigazione non accolta.

in questo caso sarei punito con la pena fino a un anno e sei mesi, non perché ho istigato all'omicidio, ma perché ho istigato al massimo dell'atto di discriminazione nei confronti del senatore Malan, non in quanto senatore, ma in quanto di religione valdese. Questo è il punto in discussione. Si potrà dire che l'istigazione deve avere delle connotazioni per essere apprezzabile penalmente: non può essere solo un dire fra due persone, anche se l'istigazione è in genere l'atto che uno compie verso un'altra persona.

viene condizionata al fatto che l'istigazione sia tale da cagionare un concreto pericolo, automaticamente per le ipotesi di cui alle lettere *a)* e il cagionare il concreto pericolo non è più richiesto, quindi è sufficiente una mera istigazione, il mero fatto verbale di compiere qualsivoglia tipo di atto di discriminazione verso una persona, perché di religione diversa, di etnia diversa, di colore diverso e quant'altro, per avere una punibilità. che un fatto assolutamente interno alla sfera privatistica, che di per sé non assume rilevanza penale per tutti i delitti anche i più gravi, verrebbe ad assumere rilevanza.

di processi in corso, al di là dell'affermazione non ne riesce ad indicare alcuno. Inoltre, quand'anche vi fosse un processo in corso perché privatamente Tizio, all'interno di un salotto, ha invitato Caio a commettere un atto di discriminazione, trovereste voi giusto questo,

per cercare di rendere questa norma sintonica al sistema che, ripeto, non punisce la mera istigazione se non accolta. Avevo parlato di un convitato di pietra. Io non ho timore. Perché l'onorevole Ferranti non ha detto le stesse cose quando questo provvedimento è giunto alla Camera? Perché, quand'è giunto alla Camera, in Commissione non ha modificato il termine «pubblicamente»? Non era forse all'epoca ugualmente esistente il pericolo del venir meno di tanti procedimenti penali? Diciamoci le cose come stanno.

che il Senato ancora esiste e non è stato abolito? Come faranno oggi i colleghi della Commissione giustizia del Partito Democratico, che hanno votato entusiasticamente l'inserimento del termine «pubblicamente» su un emendamento presentato dalla relatrice,

Certo lo potrete fare, ma allora, senatore Zanda, forse non sarà suo costume seguire i *Diktat* del convitato di pietra, ma, se dovessimo assistere a qualcosa del genere, sarà - ahimè - costume di appartenenti al suo partito. un'ultima cosa. La Costituzione assegna piena autonomia legislativa alle due Camere,

che il Presidente della Commissione giustizia della Camera, al di là dei toni usati nei confronti di quel galantuomo del senatore Caliendo, abbia potuto fare l'intervanto che ha svolto, affermando senza dati di fatto che l'inserimento del termine «pubblicamente» faceva venir meno una serie di processi ed era ispirato a chissà quale recondita e non dicibile ragione. Cercate di capire che le norme penali si ancorano alla libertà personale. Cercate di capire la cosa più semplice di questo mondo: la giustizia non bussa sempre alla porta del vicino, ma può venire a bussare a casa vostra, e quando busserà - se busserà - a casa vostra (non ve lo auguro), vi renderete conto dei guasti che state combinando con norme di questo genere

Riteniamo che non si debbano ravvisare ipotesi, che potrebbero eventualmente assurgere alla fattispecie di reati di opinione,

possa essere utile, opportuno e necessario affinché si possa ridiscutere di una norma che - ripetiamo - già di per sé è complessa, ma che in questa maniera riuscivamo a contemperare.

senatore Zanda, mi permetta, siamo in Senato - alla vergogna che questo Senato sta compiendo, con l'aggravante che è la seconda o la terza volta che sconfessa se stesso. Senato non fa passare questo subemendamento, come accadde già con l'omicidio stradale, il Senato voterà contro una sua deliberazione, assunta in Assemblea dopo un dibattito serrato, su questioni che avevano trovato unanimità. Oggi, se viene bocciato questo subemendamento sull'avverbio «pubblicamente», è il Senato che rimangia le sue stesse dichiarazioni, quindi nega, visto che siamo in tema di negazionismo, un'azione che aveva portato convintamente a circoscrivere la possibilità del reato.

e sarebbe, in caso di guerra, «dirigere deliberatamente attacchi contro proprietà civili, e cioè proprietà che non siano obiettivi militari».

hanno dichiarato che lo Stato d'Israele è razzista e che compie pulizia etniche. Quindi, questa fattispecie che noi richiamiamo si inserisce all'interno di un discorso nel quale queste azioni, se vengono negate, rientrano nella fattispecie

però c'è l'aggravante se la propaganda diffonde la mia idea. Una cosa è l'istigazione, su cui giustamente più colleghi si sono richiamati, ma noi non

tutta la questione aperta del nostro colonialismo a partire da Giolitti. Non era l'Italia fascista quella che intervenne in Libia e si macchiò sicuramente di delitti, ma si può difendere la politica italiana di quell'epoca, che probabilmente era fondata tutta sulla concezione di una supremazia etnica? Purtroppo la storia del Risorgimento era questa. Anche i piemontesi

«Pubblicamente» è il minimo che si possa mettere per dare un senso a questa norma. Quindi, noi voteremo convintamente a favore di questo emendamento.

nella Città metropolitana di Napoli.

Volevo precisare una cosa. Senatore Compagna, quando ho utilizzato l'aggettivo «compilativo», non avevo alcun intento denigratorio nei confronti di chi aveva presentato quell'emendamento.

Prendo atto, sulla base delle parole del Sottosegretario, che l'indicazione «in modo che derivi concreto pericolo» sia una soluzione mediana. A dire la verità, signor Sottosegretario, non è una soluzione mediana. Ho già citato la sentenza della Corte costituzionale del 1970, in cui sostanzialmente si dice che l'istigazione pubblica può essere punita, a condizione che sia a condizione che sia tale da cagionare un concreto pericolo. Stiamo dunque dicendo, in modo diverso, la stessa identica cosa. Comunque sia, a me va bene: diciamo che è una soluzione mediana. In virtù di questa soluzione mediana, chi istiga, fondandosi sulla Shoah, a compiere atti di discriminazione o quant'altro, in modo da cagionare pericolo, è punito da due a sei anni. Perché una analoga soluzione mediana non si può scegliere anche per l'istigazione nelle altre due ipotesi base di reato? Perché per le altre due ipotesi base di reato si deve punire un'istigazione *tout anche priva di qualsiasi capacità di creare un concreto pericolo di diffusività? Perché questo lo vorrei comprendere da voi!

a commettere un atto di discriminazione nei confronti del senatore Malan, di religione valdese, vengo punito anche se questa istigazione non è tale da cagionare alcun pericolo? pericolo? Se è una soluzione mediana, signor Sottosegretario, se è una soluzione di buon senso ‑ e abbiamo già detto che non lo è, ma ove mai lo dovesse essere - non sarebbe allora ugualmente mediano inserire nelle altre due ipotesi base di reato questa postilla, questa qualificazione dell'istigazione, in modo da cagionare concreto pericolo o, se si vuole, in modo da cagionare pericolo, quindi parlando di pericolo del pericolo, con un'ampia discrezionalità da parte del giudice? Come potete voi consentire il permanere in vita di una norma, che conferisce apprezzabilità penale, in termini anche pesanti, fino a quattro anni, come recita la lettera *b),* quando quella istigazione rimane un fatto

tenendo presente che la sanzione penale va a comprimere la libertà personale dei soggetti e che, per comprimere la libertà personale dei cittadini, forse sarebbe necessario che i fatti abbiano realmente una loro lesività. ai cittadini, a quei cittadini cui spesso si richiama il Movimento 5 stelle. Non vi rendete conto, voi che fatte tanta opposizione a parole nei confronti del Partito Democratico,

in modo da consentire un'unicità di trattamento ai diversi cittadini in ordine a comportamenti che vengono considerati penalmente apprezzabili. Come potete non rendervi conto del fatto che la circostanza aggravante aumenta la sanzione con riferimento ad una circostanza che aggrava il fatto base, non modificando il fatto base, non modificando l'istigazione semplice in un'istigazione che crea concreto pericolo? Ma, quando arriveremo a quell'emendamento, vi rivolgerò cortesemente e nuovamente l'invito. Signora Presidente, vedo che il collega Palma, giustamente, si preoccupa di circoscrivere l'istigazione in maniera tale che essa debba avvenire pubblicamente e non sia considerato istigazione anche un colloquio fra due persone, cioè un fatto privato. Io mi preoccupo di questo e voterò a favore dell'emendamento. Ma mi preoccupo di più del fatto che l'idea,

è in sintonia con una certa storia; evidentemente gli anni passano, ma l'idiosincrasia per la libertà e per le opinioni degli altri rimane, solo che, una volta, si applicava con le tragedie della storia, adesso si applica con battute che forse andrebbero bene per Checco Zalone. Ora, poiché molte persone ci ascoltano (non è vero che i lavori del Parlamento non siano seguiti)

e se pubblico questo libro, c'è un concreto pericolo di diffusione? Ma va! Le idee che vengono scritte sono sottoposte ad un concreto pericolo di diffusione. che io le diffonda; il solo fatto che io le pubblichi o che scriva un articolo mi costa fino a sei anni di carcere. Persone che ci ascoltate da casa, le cose che ho detto prima e che dico adesso nessuno le contesta. Nessuno spiega perché si debba far passare questa vergogna di paragonare l'Olocausto ad altre migliaia di casi, alcuni dei quali bagattellari rispetto a quella tragica esperienza storica. Se vi leggo le cose che vi ho letto - suggerisco a Checco Zalone di riprenderle come *gag* di un suo spettacolo - qualcuno forse può dirmi che non sono scritte così? Silenzio, perché non lo potete smentire; è agli atti: sono le cose che qualcuno, nella notte, ha scritto, scavalcando l'intera Commissione e facendo trovare tutta l'Assemblea in un grande imbarazzo. Infatti, chi ha una qualche esperienza di Parlamento capisce benissimo che le cose che si stanno dicendo sono talmente ovvie che vedo la sofferenza nel volto dei colleghi, soprattutto dopo lo scriteriato intervento della rappresentante del Governo, che è entrata a piedi pari a dare un parere favorevole quando in Commissione, viceversa, non si era mai neanche sognata di proporre soluzioni di questo tipo. Anche questo è uno strano rapporto Governo-Parlamento. Sulle unioni civili si sono rivolti alla Commissione dicendo che il Governo

anzi, con il silenzio ha avallato la soluzione che era stata presa sostanzialmente all'unanimità dalla Commissione, con qualche dissenso, compreso il mio - e questa mattina il Sottosegretario dà parere favorevole all'emendamento notturno, quello di Checco Zalone:

e quando pone problemi sistematici del codice penale, mi meraviglia la vostra sovrana indifferenza. Certo, tanto saranno i cittadini a finire sotto processo; a voi cosa interessa? Finché non toccherà a qualcuno

questo emendamento, tornando a insistere che non è risolutivo - perché non risolve il problema delle idee - ma almeno fa capire che un'istigazione per essere colpita così duramente quantomeno deve avvenire in maniera pubblica.

Vero è che l'atteggiamento avuto dalla Camera nell'eliminare l'avverbio «pubblicamente» - dopo che qui in Senato è stato votato forse all'unanimità, o comunque

quando proviene, non già da un semplice deputato, ma da chi ha la responsabilità di governare la Commissione giustizia della Camera. Perché dico falso problema? Perché il il significato dell'espressione «pubblicamente» ce lo indica il codice penale all'articolo 266, quando dice espressamente che, agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso «in luogo pubblico o aperto al pubblico

questo, nel momento in cui il senatore D'Ascola, presidente della Commissione giustizia di questo Senato, questo Senato, con il proprio emendamento dice testualmente «ovvero l'istigazione e l'incitamento commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione», è chiaro che questo pericolo di diffusione va rapportato «pubblicamente». Ecco perché io dico che sostanzialmente non vi è alcuna differenza. È soltanto un modo per meglio chiarire e - ahimè, checché ne pensino alla Camera - per meglio e ancor oltre ribadire la nostra esigenza che l'istigazione debba avvenire pubblicamente, ovvero anche soltanto in modo un concreto pericolo di diffusione. È evidente l'esempio che ha fatto il senatore Giovanardi: nel momento in cui pubblico una tesi e la diffondo, è chiaro che si è realizzato quel concreto pericolo di diffusione.

effimero. Ho apprezzato lo sforzo del senatore D'Ascola nell'aver immaginato una soluzione che, se mi consentite, definirei un po' come l'uovo di Colombo:

di dichiarazione di voto, non mancherò di essere ancora più severamente critico rispetto a chi ritiene di condizionare, anche esercitando il proprio ruolo di responsabilità

a ciascuno sia lasciata la sensibilità di decidere sulla base della propria coscienza, della propria storia e delle proprie considerazioni che sul tema si possono fare, e sono tante. **Saluto

si persegue l'effetto di contenimento del danno sotto il profilo della coerenza dell'impianto penalistico del nostro ordinamento.

da parte del Senato era una soluzione mediana tra la Camera e il Senato non ci ha convinto; in primo luogo, perché una soluzione mediana non può prescindere dal dibattito che c'era stato in Assemblea. Non vi è stato un solo intervento, un solo accenno alla inopportunità del «pubblicamente». Ma una soluzione mediana meno ancora può essere quella che riconduce, poi, il giudizio di apprezzabilità di un comportamento alle circostanze più casuali. Da questo punto di vista, le ragioni per le quali

che non vi siano, invece, ragioni a favore del subemendamento da parte di coloro che, invece, non escludono di votare a favore dell'emendamento D'Ascola. Questo è sorprendente ma non induce noi a un voto diverso dal voto favorevole all'emendamento 1.401/3.

si sia sbagliato nel votare perché ha votato contro il subemendamento dopo aver sviluppato un ragionamento - se non ho mal compreso - tutto a suo favore. Cosa dice il senatore Falanga? il problema che si pone è un falso problema. È chiaro, infatti, che l'istigazione deve cagionare pericolo e poi aggiunge che l'istigazione non può che essere pubblica, perché così afferma l'articolo 414 Io sono assolutamente d'accordo con il senatore Falanga: l'istigazione, per essere apprezzabile penalmente, non può essere un'istigazione non accolta o commessa solo in sede privata. esattamente d'accordo con lei, senatore Falanga, ed è esattamente quello che noi vogliamo. Vogliamo che si chiarifichi alle lettere di riferimento ciò che il relatore e il Presidente hanno inteso chiarificare al terzo comma: che anche l'istigazione delle ipotesi base sia una istigazione penalmente apprezzabile e quindi o commessa pubblicamente o, se si vuole, nella fantomatica ipotesi mediana, commessa in modo tale da cagionare concretamente il pericolo di diffusione. Non chiediamo nient'altro. Però vi pongo un problema: nell'eventualità in cui voi doveste votare contro questo emendamento e principalmente contro il successivo, che ripete per la lettera *b)* la stessa formula indicata dal presidente D'Ascola nel suo emendamento, vi trovereste per l'ipotesi segnalata dal senatore D'Ascola di fronte a un altro tipo di reato,

Invece, per la ipotesi del senatore D'Ascola, questa istigazione deve essere tale da cagionare un concreto pericolo. Quindi ci troviamo di fronte a una fattispecie del tutto diversa. Voi continuerete a votare contro questi emendamenti, ma consentirete a noi di continuare a sostenere le nostre tesi.

per questi fatti non esistono e molto probabilmente non esisteranno, non vi saranno modo e motivo di interessare la Corte costituzionale. Ma se non esistono e non esisteranno, perché l'onorevole Ferranti afferma che l'inserimento del termine pubblicamente o similare fa venire meno non so quante centinaia di processi? Se non esistono, non esistono. Quindi voi farete un'operazione in ossequio a chi realmente comanda, ma farete un'operazione sotto il profilo tecnico assolutamente sbagliata.

visto che le cose hanno un'attinenza con la libertà di opinione. È una verifica che sto facendo quindi non sono ancora in grado di confermare, però è meglio essere prudenti quando si tratta di libertà di parola. Ho voluto approfondire di nuovo il combinato disposto, perché dico anche ai colleghi che hanno seguito la questione in Commissione che per comprendere quello che stiamo facendo non basta avere il testo della legge approvata in Commissione.

una persona per capire su che base può essere incriminata, non basta che legga la legge, ma deve leggere la norma originaria e poi tentare di fare il collegamento tra quanto previsto nella norma originaria e l'aggravante prevista nel nostro caso esame. Cosa dice la legge originaria alla lettera *a)*? Che viene punito con la reclusione fino a un anno e sei mesi

la diffusione, la divulgazione, la propagazione, il proselitismo l'apostolato delle idee. Quando si parla della propaganda delle idee, è evidente che dentro la propaganda c'è la diffusione, non è che ci sia il pericolo concreto di diffusione della propaganda: è *in re ipsa*. Quello che è stato scritto sul testo è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Ma voi direte attenzione i sei anni di condanna li prendi se richiami questioni che hanno a che fare con le

stampa, ha condannato le pratiche di Israele sulle terre palestinesi occupate, accusandolo di complicità in segregazione razziale e pulizia etnica. Era forse uno che passava per strada? No, era stato nominato relatore su queste

commette pulizie etniche e odio razziale proprio mentre interviene nelle fattispecie che loro definiscono crimini di guerra. Dopo di che, altro che Olocausto, caro Zanda!

mettendo il Senato e i membri della Commissione davanti a un nuovo testo che peggiora grandemente la situazione. Pertanto, anche io direi basta, torniamo in Commissione, perché stiamo scrivendo una norma che non ha senso; poiché così non accade, è chiaro che emendamento per emendamento sarà nostro dovere fare l'approfondimento e, se volete, *repetita iuvant*, per farlo capire nel silenzio. Capisco

se dovesse passare la questione che sto verificando, possa trovarsi incriminato per una questione che è semplicemente l'espressione di un'idea su decine di migliaia di casi che avvengono in tutto il mondo.

Tra le altre cose, gran parte di loro fa parte della comunità ebraica e, quindi, avrebbe dovuto essere anche interessato, ma quegli storici hanno sottolineato il pericolo di un testo che, invece di stigmatizzare l'Olocausto, si trasforma in un atto liberticida. Per queste ragioni voteremo a favore del subemendamento

non esiste un'istigazione privata e in tutti gli articoli in cui si parla di istigazione è ripetuto l'avverbio «pubblicamente». Vi rendete conto che se non lo inseriamo, con la bocciatura del subemendamento precedente, che tra l'altro era identico all'emendamento a

diversa? Se volete recuperare, questa è allora l'unica possibilità che abbiamo, altrimenti ci troveremo di fronte a un provvedimento di difficile e difforme e difforme applicazione e con contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione se il Parlamento abbia voluto introdurre una nuova fattispecie di reato o un'aggravante. Non si riesce a far comprendere che quindi è un fatto tecnico.

quando dicevo che bisognava introdurre le valutazioni e voi avete detto di no? La Cassazione è dovuta intervenire a sezioni unite. Abbiamo avuto sentenze della Cassazione che hanno assolto per il falso valutativo e abbiamo avuto sentenze della Cassazione che hanno condannato e ci è voluta una sentenza delle sezioni unite per arrivare alla continuità normativa, semplicemente perché, anche in quella occasione, la maggioranza volle votare per una questione di principio e non per il merito del provvedimento.

perché, proprio con gli argomenti che richiamava adesso il senatore Caliendo, se si dovrà pronunziare in favore dell'emendamento 1.401, anche questo subemendamento di Caliendo, in assoluta coerenza con il precedente di Palma, serve per ridurre il danno, per ridare omogeneità, se non coerenza, al nostro ordinamento penalistico, o ancora, sotto un profilo costituzionale, alla valutazione di ciò che deve essere penale e di ciò che assolutamente non deve essere penale. Che la discussione avesse questo come centro lo avevamo avvertito proprio in occasione del passaggio alla Camera.

Che vuol dire il richiamo alle giurisdizioni internazionali? Che bersaglio ha se non il solito, lo stesso del 25 aprile? Lo Stato d'Israele, colpevole ontologicamente di razzismo. Da qui discende la necessità di un riferimento normativo nell'ordinamento italiano per adire la giurisdizione internazionale. Con profondo merito del presidente D'Ascola e di tutti quelli che hanno lavorato in Commissione giustizia ci era giunto un testo che cancellava queste corsie privilegiate di antisemitismo dettato da antisionismo. Se ho diritto anche io a fare una citazione, è quella di un collega prestigioso, il senatore a vita Giorgio Napolitano. Rimettere in gioco inopinatamente quel testo, cancellando il «pubblicamente», crea un equivoco che l'ordinamento si trascinerà a lungo e colpisce la libertà delle libertà: la libertà di opinione. Noi voteremo a favore del subemendamento 1.401/5, memori anche di una vecchia battuta. Luigi Einaudi diceva che la migliore legge sulla libertà di opinione è nessuna libertà di opinione. Era un dubbio al quale eravamo disposti a rinunciare, ma quando invece vediamo che subdolamente, senza neanche giustificarlo ad alta voce in questa Aula, dai membri dell'altro lato dell'emiciclo viene cancellato il «pubblicamente», la nostra nostalgia per il «pubblicamente» data quarantotto ore, ma è fortissima. Di qui il voto favorevole all'emendamento 1.401/5.

la cultura sia un passaggio fondamentale nel nostro Paese per riuscire a risolvere questa problematica. Solo la cultura potrà risolvere un problema che riguarda proprio la discriminazione

non si confondano cose storicamente accertate e sacre, con delle bagattelle. Quindi, la nostra proposta è quella di mantenere fermo l'articolo 6 della Convenzione internazionale, laddove parla di genocidio e di Shoah, ma di espungere gli altri due articoli, che

«distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala illegalmente e arbitrariamente; deportazione, trasferimento o detenzione illegale; dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità; lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi danni all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti». Non so se vi rendete conto: vengono danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti;

Vi rendete conto di tutte queste cose che vi ho letto - ad esempio anche: «distruggere o confiscare beni del nemico, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalla necessità della guerra; violare la dignità delle persone, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti» - sono esattamente tutte le accuse che vengono mosse a Tsahal, all'esercito israeliano, e a Israele, accusandolo di fare pulizia etnica e di avere un atteggiamento razzista? Vi rendete conto che queste fattispecie sono proprio quelle

è chiaro che in questo caso il numero legale c'è stato perché gli originali richiedenti erano in numero cospicuo. Ma ella ha il dovere di verificare se gli originali richiedenti sono presenti in Aula oppure no, ancorché non votanti.

sottoposto ad una costante verifica, perché diversamente si altera il significato della nostra presenza in Aula. Penso che anche coloro che sono convinti della bontà del fatto che i nostri voti debbano essere prevalentemente espressi con il sistema elettronico siano d'accordo su questo principio. Altrimenti sono costretto Altrimenti sono costretto a chiederle di rivedere la prassi in seno alla Giunta per il Regolamento e di revocare l'autorizzazione a che la richiesta di voto elettronico possa valere per un numero "x" di

di ritornare alla prassi precedente, perché questa è un'innovazione dell'attuale legislatura. Il voto elettronico, come dice il nostro Regolamento, deve essere richiesto volta per volta così da avere effettivamente la certezza che il richiedente sia in Aula. Altrimenti la Presidenza, non dico ad ogni votazione, ma soprattutto quando si verifica un evidente calo di presenza in Aula, deve verificare se gli originali richiedenti sono presenti.

il voto elettronico ad inizio di seduta e poi mi allontano. Lei dovrebbe far rimuovere le tessere e quelle tessere non dovrebbero essere abilitate a

diventa veramente una farsa se dobbiamo dire che dobbiamo togliere la tessera e far risultare che non siamo presenti.

D'altra parte, mi pare anche molto sensato e approfondito quanto detto dal senatore D'Alì, è evidente che, al di là della prassi, è difficile in generale continuare i lavori sulla presunzione di una situazione che i fatti hanno modificato. Signora Presidente, credo che questo sia un classico caso in cui gli equilibri instabili della Giunta per il Regolamento non dovrebbero impedirci di riunirla e di portare in il quesito intorno a una situazione reale che si è verificata in Assemblea. Non c'è bisogno di farlo immediatamente. Occorre, però, che rimanga a verbale il fatto che questa situazione è accaduta

la richiesta che, al più presto e non in questo momento, la Giunta per il Regolamento prenda in considerazione la situazione e arrivi a una determinazione di fronte al fatto che lei non poteva giudicare diversamente, ma che il senatore D'Alì

Presidente, mi perdoni, ma relativamente al concetto di prassi, vorrei far notare che qualunque prassi può instaurarsi in qualunque momento e diventare tale solamente dopo un certo numero di iterazioni dello stesso principio.

Faremo una verifica per vedere chi è presente all'interno dell'Aula e rifacciamo la votazione», per onore di correttezza. Segretari, né i Questori, né altri hanno eccepito alcunché. Quanto alla prassi, tanto per essere precisi, io avevo detto che si instaura come consuetudine e questa è codificata anche da un parere della Giunta per il Regolamento. In considerazione

Siamo agli interventi di seduta, senatore Giovanardi. Io ho proclamato l'esito della votazione, dicendo che si votava la prima parte, fino alle parole: «dall'articolo 6», e, quindi, era precluso tutto il resto, perché nel più sta il meno. Se si vota e si respinge la prima parte, tutto il resto non sta in piedi e, quindi,

Presidente, intervengo, se il senatore Giovanardi permette. Oggi si celebra la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro voluta dalla OIL, Organizzazione internazionale del lavoro, agenzia dell'ONU. Quest'anno detta celebrazione è dedicata allo *stress* lavoro-correlato e ai rischi psicosociali. Sotto questo profilo, è utile ricordare che l'articolo 28 del testo unico sulla sicurezza impone a tutti i datori di lavoro di valutare lo *stress* lavoro-correlato, cioè il rapporto tra l'organizzazione dell'attività e la salute, intesa quale stato di completo benessere fisico. Presidente, onorevoli colleghi, è utile ricordare altresì che oggi si celebra la Giornata mondiale dedicata alle vittime dell'amianto. Secondo un rapporto dell'Organizzazione mondiale della sanità, sono circa 15.000 le persone che ogni anno in Europa perdono la vita a causa di patologie amianto-correlate e sono 21.000 i casi registrati in Italia dal 1993 al 2012, di cui il 70 per cento presenta una diagnosi certa, probabile o possibile di esposizione professionale all'amianto, e solo l'1,6 attribuibili a una causa extralavorativa. Signora Presidente, molto è stato fatto da quando nel 1992, con la legge n. 257, si è bandito l'amianto in Italia, ma riteniamo che ancora molto sia da fare e che il tema e la sua rilevanza sociale, di giustizia, di salute e di ambiente, imponga l'assunzione di responsabilità per trovare una soluzione definitiva da parte del Parlamento e di tutte le forze politiche.

fu ancora una volta profeta sul caso Lande srl, questa volta, e su supposti appalti pubblici che favorirebbero i casalesi. All'epoca la questione fu sollevata dal deputato al ministro Franceschini in ordine al secondo filone d'inchiesta su Pompei, per corruzione e turbativa d'asta, aggravata dal metodo camorristico a favore del clan Zagaria dei casalesi, da parte appunto dell'allora dell'amministratore Si chiedeva, allora, nel *question time*, di attivare ispezioni e controlli sui numerosissimi appalti pubblici della Lande, che sono in tutta Italia, ma Franceschini scivolò, minimizzò e glissò. Il deputato Gallo, però, non risparmiò di dire al Ministro che lo avremmo ritenuto responsabile se in futuro altre inchieste su questa società si fossero dovute presentare. E così è stato. Due giorni fa il PD è stato travolto da una nuova inchiesta che coinvolge la società in questione, e che ha portato in carcere ben nove persone, tra cui l'ex sindaco di Santa Maria Capua Vetere Di Muro, di una lista sostenuta dal PD, e il Presidente del PD campano Stefano Graziano, per un appalto pubblico per il recupero del palazzo Teti, immobile confiscato alla camorra. antimafia di Napoli, la gara sarebbe stata vinta da un raggruppamento di imprese vicine al clan Zagaria (di nuovo), tra cui ritroviamo la società Lande. Graziano, che è consigliere regionale di maggioranza, da intercettazioni telefoniche sarebbe stato eletto grazie ai voti della camorra, a mezzo dell'imprenditore di Casapesenna Alessandro Zagaria, Graziano si dimetta dal Consiglio regionale, come è stato già richiesto dal nostro portavoce regionale Malerba, e che si attivino tutte le ispezioni e i controlli necessari sui numerosissimi importanti appalti pubblici vinti della società Lande in tutta Italia, che - ricordiamo - è quasi sempre ovunque presente nelle inchieste che ci sono state negli ultimi dieci anni per infrastrutture e lavori pubblici in tutta Italia, da Alessandria, a Pompei, al G8 della Maddalena, ai lavori per l'Alta velocità, ai lavori per l'Unità d'Italia, fino fino alla recentissima inchiesta sulla Total della procura di Potenza. La Lande c'è sempre.

attuale, stradiscussa, ma non risolta. È una questione sulla quale il legislatore ha agito, ma non efficacemente. Ad esempio, la legge n. 175 del 2010, la cosiddetta legge Lazzati,

oltre a tutta un'altra serie di «se» e di «ma». Immaginate un mafioso fare campagna elettorale affiggendo manifesti o facendo volantinaggio? Nell'aprile 2013 è stato presentato, a prima firma del senatore Molinari, il disegno di legge n. 455, volto a eliminare tutte le limitazioni che avevano reso inefficace la legge Lazzati.

Chiedo alla maggioranza di passare dalle parole ai fatti per affrontare realmente il tema di liberare tutta la politica da rapporti opachi ma oscenamente vantaggiosi con la criminalità organizzata. Se non si allontana la mafia dalla Repubblica, diventa insopportabilmente ipocrita celebrare gli eroi che, isolati, si contrappongono alle mafie. Questo è fondamentale. È una scelta fondamentale che va presa presto, per superare le contrapposizioni da comunicato stampa e fare quello che il legislatore deve fare: buone leggi.

Grazie,